Onorevoli colleghi, nella serata di ieri, all'età di 83 anni, si è spento nella sua casa romana, dopo una lunga malattia, l'editore Carlo Caracciolo. Tratteggiare la biografia di quest'uomo, elegante e coraggioso, innamorato della vita e della professione di editore, significa ripercorrere, in qualche modo, la storia del giornalismo italiano dell'ultimo mezzo secolo. Dopo l'esperienza partigiana in Val d'Ossola, la laurea in giurisprudenza a Roma e il perfezionamento ad Harvard, si era dedicato all'editoria, fondando una piccola casa editrice di riviste tecniche rivolte al mondo dell'industria. Nel 1955, assieme a quell'altra straordinaria figura dell'imprenditoria italiana che fu Adriano Olivetti, aveva partecipato alla fondazione del settimanale «L'Espresso», per poi assumere, l'anno successivo, il ruolo di azionista di maggioranza. Nel 1976, nel momento in cui la gestione del settimanale iniziava a consolidarsi, non esitò a tornare a rischiare, ponendo le sue straordinarie doti di audacia imprenditoriale e di coraggio civile al servizio dell'ambizioso obiettivo di costituire un grande quotidiano nazionale. Il gruppo editoriale da lui diretto fu allora tra i protagonisti della fondazione del quotidiano «la Repubblica». Questa propensione al rischio, in nome della valorizzazione della professione giornalistica e di una significativa presenza civile e culturale nella società, lo condusse ad intervenire, fino agli ultimi anni della sua vita, in imprese editoriali che apparivano ai più assai difficili, com'è avvenuto nel 2007, per il salvataggio del quotidiano francese «*Libération*». Quest'ultima impresa gli valse, presso la stampa d'Oltralpe, l'appellativo dell'«uomo che non ama veder morire i giornali». Non si trattava soltanto di acume imprenditoriale: per Carlo Caracciolo l'editoria costituiva un poderoso strumento di impegno civile e culturale, il canale attraverso il quale esprimere una nobile ed irrefrenabile passione politica, vissuta però con lo stile e la misura che l'hanno sempre contraddistinto. Con la sua scomparsa, l'Italia perde un editore vero, tra i pochi in grado di coniugare cultura e mercato, progetti commerciali e impegno politico. A nome di tutta l'Assemblea e mio personale, esprimo quindi il più sentito cordoglio e una viva partecipazione al dolore della sua famiglia e a quello dei giornalisti e dei dipendenti del gruppo editoriale l'«Espresso» e delle numerose società editoriali nelle quali svolse un ruolo da protagonista. Invito pertanto tutti i colleghi ad osservare un minuto di raccoglimento.

Signor Presidente, colleghi senatori, oggi l'Aula ricorda Carlo Caracciolo, definito da tutti l'ultimo grande editore puro esistente nel nostro Paese. Storico fondatore del gruppo editoriale «L'Espresso» e del quotidiano «la Repubblica», Caracciolo decise di dedicare tutta la sua vita alla causa dell'informazione. Egli stesso definiva il suo lavoro come l'assolvimento di un compito civile, convinto del ruolo imprescindibile del buon giornalismo per lo sviluppo della vita democratica e la crescita della società. Si è spento ieri, a 83 anni, dopo una lunga malattia e dopo aver attraversato da protagonista tante importanti fasi della storia del nostro Paese. Dapprima le battaglie antifasciste, da partigiano in Val d'Ossola, poi, negli anni Cinquanta, l'inizio di quella che sarebbe stata

la specializzazione ad Harvard, l'incontro con l'imprenditore Olivetti, le prime riviste tecniche, il settimanale «L'Espresso», fin quando nel 1976 divenne presidente e amministratore delegato della società editrice «la Repubblica», che iniziò le pubblicazioni del quotidiano diretto da Eugenio Scalfari. Nel racconto dei fatti che hanno cambiato la storia del nostro Paese, dal rapimento di Aldo Moro a Tangentopoli, passando per le battaglie civili, Carlo Caracciolo riuscì a far diventare il suo quotidiano un indispensabile punto di riferimento culturale per i lettori, al di là del suo credo politico di cui non ha mai fatto mistero. Chi ha avuto l'opportunità di accompagnarlo nel suo percorso di vita lo ha descritto come un uomo di grande curiosità intellettuale, animato da passione vera per la professione, fine, spiritoso e sincero. Ed era soprattutto un grande amante dei quotidiani, che non si limitava a leggere, ma che ritagliava, conservava e di cui cercava l'anima e il senso. Tutte attitudini queste non solo da vero editore, ma anche da buon giornalista. Furono molti quelli cui diede coraggiosamente fiducia fin da giovanissimi e che, assieme a molte grandi firme, contribuirono al successo delle sue creature editoriali. È anche per questo spiccato amore per il giornalismo a tutto tondo che decise, nel 2007, di acquistare quote del giornale francese «*Libération*» per salvarlo dal dissesto finanziario. Negli ultimi giorni, spesi a combattere il brutto male che lo affliggeva, sembrava fosse molto amareggiato dalla situazione politica italiana e dal fallimento degli ideali in cui era cresciuto. Il protagonismo e l'avidità sempre più presenti nella nostra società, se confrontate con la sua figura sobria, forte e concreta, ci lasciano un velo di nostalgia e un grande vuoto. Con Carlo Caracciolo l'Italia perde un uomo vero, un maestro e un padre dell'editoria. Resta la speranza che il suo insegnamento diventi un modello da seguire per tanti giovani e che «l'ultimo Editore» trovi degni e appassionati successori.

dovesse commemorare un personaggio sì di grande rilievo, ma estraneo al mondo delle Aule parlamentari. La spiegazione sta senz'altro nel fatto che, al di là della sua dimensione di gran signore, di persona intelligente, colta e intraprendente nel mondo degli affari, Caracciolo ha rappresentato, forse nel più elegante dei modi, quello che siamo abituati a chiamare il quarto potere. Quanto questo quarto potere sia imbarazzante nel mondo della politica italiana lo ricorda bene Umberto Eco in una traccia comparsa riportando che Caracciolo, proprietario di case editrici come Etas Kompass, Bompiani, Sonzogno, Adelphi, Boringhieri e Publikompass, diventò involontariamente il bersaglio di un ricatto sul cognato Giovanni Agnelli. Caracciolo veniva ricattato via Agnelli e (cito sempre dalla sua autobiografia, anche se si tratta di cose che ricordo benissimo per conto mio) Fanfani aveva preso a dire che se Caracciolo non avesse ceduto le sue quote dell'Espresso a persona gradita alla segreteria democristiana, il governo avrebbe bloccato l'aumento del prezzo delle automobili». Curioso esempio di interventismo; non so se fosse lecito, ma si poteva pensare. Caracciolo aveva dovuto scegliere con il coltello alla gola se stare con le sue case editrici e mollare l'Espresso, o tenersi l'Espresso e interrompere ogni rapporto con le società legate alla FIAT. Aggiunge Umberto Eco: «È mio parere che il gruppo delle case editrici rappresentasse il boccone più grosso, ma il "principe" non ha avuto esitazioni. Ha mollato l'editoria e si è tenuto l'espresso. Non era stata una scelta facile e non fosse altro che per questo Caracciolo andrà ricordato come un editore che ha pagato per per difendere la libertà di stampa». Sarebbe ipocrisia tacere che, dopo questo episodio tutto sommato veniale del sottogoverno democristiano, l'impresa editoriale di Caracciolo è stata sottoposta a ben altra tensione.

La guerra di Segrate è presto riassunta. Fu il tentativo da parte di Bettino Craxi di impadronirsi, tramite le finanze di Berlusconi, del giornale a lui più inviso e del gruppo editoriale più insidioso per la sua politica. Una cosa di questo tipo va ricordata anche perché in quella storia si è verificato, con il tempo, un mutamento di ruolo. Nel momento in cui agiva nella guerra di Segrate, Berlusconi era poco più che un caudatario di seconda fila di Bettino Craxi:

Purtroppo, con il tempo, si è visto che Berlusconi aveva anche una capacità propria di agire in proprio. Una volta affrancato dalla protezione di Craxi, ha esercitato un'influenza molto più stringente e molto più invasiva ed incisiva di quella che aveva esercitato al tempo della guerra di Segrate. Che dire? Traiamo da questa storia molti insegnamenti. Uno, di sicuro, può essere scolpito nelle nostre menti. Il fatto che il quarto potere della stampa ha subito la minaccia dell'unione tra quarto e quinto potere nella persona di Berlusconi protetto da Bettino Craxi. Ma traiamo anche un altro insegnamento: che per il bene della democrazia e del dibattito pubblico in Italia sarebbe molto più sensato, molto più rigoroso e significativo se il quarto ed il quinto potere fossero rigorosamente separati tra di loro e, soprattutto, se il quarto e il quinto potere fossero

La scomparsa di Carlo Caracciolo rappresenta sicuramente una perdita per il mondo della cultura, la perdita di un uomo che ha saputo caratterizzare la propria vita con l'impegno antifascista

Ebbe intuizioni ed ebbe anche un grande coraggio, anche quando le sue creature - specie agli esordi, agli inizi - vissero momenti di difficoltà.

Si dichiarava uomo di sinistra, ma non comunista ed era capace di onestà intellettuale e di rispetto dei ruoli. Il suo legame di parentela con Gianni Agnelli non condizionò mai le sue scelte, che lo videro sempre esprimersi in libertà e autonomia di pensiero. Due personaggi legati non solo da un intreccio familiare, ma anche da una vecchia complicità giovanile. Quindi, fu un uomo di cultura e un signore nello stile, senza fronzoli, che è stato al centro della cultura e dell'evoluzione del Paese. Impegnato per la politica, ma non in politica, condizione che gli permise di essere libero editore anche se fortemente connotato sul piano ideologico. lo sappiamo bene, viste anche le considerazioni e i diversi attacchi che il nostro movimento ha subito da quelle testate. Ma tant'è! Scompare un'altra figura fortemente impegnata sul piano civile, nella quale le passioni sapevano essere il motore per caratterizzare una vita significativa e densa di emozioni ed avvenimenti. *(Applausi dai Gruppi

ieri sera. Noi senatori saremmo ciechi se non sapessimo riconoscere lo straordinario rilievo pubblico che la nostra società ha ha assegnato agli editori, ai direttori dei giornali influenti, agli editorialisti importanti e, più in generale, a tutto il mondo dell'informazione. Quindi, nel poco tempo che ci è consentito dai nostri lavori d'Aula, credo sia giusto che oggi il Senato partecipi al lutto della famiglia Caracciolo, dell'editoriale «L'Espresso» e di tutta l'editoria italiana per la scomparsa di quello che in tanti consideriamo essere stato, nel mondo della stampa periodica e quotidiana, il nostro più grande editore del dopoguerra. Chi lo ha conosciuto sa bene quanto Caracciolo detestasse la retorica e quanto, se avesse potuto, ci avrebbe chiesto di non farne uso in queste circostanze. In poco più di cinquant'anni, partendo da un settimanale di politica, economia e cultura, «L'Espresso», per mano di Carlo Caracciolo è pian piano cresciuto nel nostro Paese un vastissimo gruppo editoriale, formato da un quotidiano nazionale, da quotidiani locali, da periodici di cultura politica, di analisi geopolitica, di ricerca scientifica, da concessionarie di pubblicità, da tipografie, da televisioni e da radio. A queste imprese - lo ha ricordato anche lei, signor Presidente - pochi anni fa Caracciolo aveva voluto aggiungere una personale partecipazione all'avventura parigina del salvataggio di «Libération»

colleghi, questa colossale opera, che insieme è stata industriale, culturale, politica e sociale, le cui vicende sono così profondamente intrecciate con la storia del nostro Paese, ha tanti autori quante sono le persone che hanno contribuito a costruirla (direttori, giornalisti, dirigenti, personale amministrativo e tecnico), ma ha avuto un solo regista, un solo ideatore e un solo padre: Carlo Caracciolo. E di lui basterebbe ricordare quello che ha saputo costruire con il suo lavoro e con le sue iniziative per assegnargli un posto d'onore nel nostro Pantheon nazionale. Ma io credo che lo si debba onorare, oltre che per il tanto che ha realizzato, per "come" ha vissuto il suo impegno di editore italiano e per "come" ha saputo proporre al Paese un nuovo modo di fare informazione. È stato già ricordato che era uno spirito libero, ricco di interessi e di curiosità e fortemente attratto dalle cose nuove. Gli piaceva tutto ciò che

ha trasformato il grande «Espresso» in un *magazine*: era un'assoluta novità per l'Italia ed ebbe in seguito tanto imitatori. Poi con il suo amico Eugenio Scalfari ha trasferito, adattandola, l'esperienza de «L'Espresso» a «la Repubblica», che sin da quando è nata ha avuto una diffusione nazionale, innovativa nel formato, nella distribuzione, nei centri stampa, la prima nell'adottare il colore, la prima nei supplementi, la prima nella diffusione abbinata quotidiano-libro. Tutto questo senza perdere mai di vista l'esigenza di un'informazione di qualità e soprattutto l'impegno civile.

era considerata da tutti un suo personale capriccio, il sogno di un visionario. Ed invece aveva ragione lui: è proprio nella realtà dei quotidiani locali che si riflettono le 100 città che costituiscono l'ossatura forte del nostro Paese. Ricordo, nella seconda metà degli anni Settanta, le sue prime mosse pionieristiche e i quotidiani di Livorno, Sassari, Pavia, Padova, Treviso, Venezia e poi tanti altri. Oggi sono 18 testate. Questo è stato il progetto innovativo di Caracciolo, un «editore puro», come si diceva una volta. Aveva un disegno chiaro in mentre e, in un Paese di improvvisatori come il nostro, l'ha messo in atto con rigore assoluto, pezzo dopo pezzo, pagina dopo pagina, impegnandosi ogni volta allo spasimo, lavorando su ogni più piccolo problema come se fosse quello decisivo. Lui diceva spesso: «Sono i piccoli fiumi a fare i grandi mari». E l'aspetto più straordinario, ciò che fa di Caracciolo un editore speciale, è la tenacia sempre lucida con cui ha lavorato per una vita alla realizzazione del suo progetto. Circostanze impreviste potevano fermarlo e ostacoli esterni potevano costringerlo a rallentare la marcia. Ma non si dava mai per vinto, ripartiva sempre e mai, mai si sentiva sconfitto: era un vero combattente. Di lui si può dire che considerava il suo mestiere di editore una missione civile e nutriva quotidianamente il suo lavoro non solo di idee nuove e di fantasia, ma anche di azioni sì coraggiose, ma mai spericolate. Con lui sapevi che una stretta di mano contava più di qualsiasi contratto. Termino ricordando il suo impegno politico, perché Caracciolo era politicamente molto impegnato. Anzi la politica è stata una parte rilevante della sua vita. Lo è stata quando, a 18 anni, ha partecipato alla guerra partigiana e lo è stata poi nella lunghissima vita di editore. Ma era troppo elegante nel pensiero ed elegante nel profondo del suo animo per trasformare il suo impegno politico in faziosità, in travisamento della realtà, in discriminazione nei confronti di chi non la pensava come lui. Era un democratico vero. L'impresa editoriale che ha compiuto è straordinaria per la vastità e la consistenza dei risultati, ma ancor di più per la qualità civile che l'ha permeata e di cui tutt'oggi è intrisa. Dietro imprese di così tanta qualità, signor Presidente, ci sono sempre uomini speciali, uomini anch'essi di grandi qualità e Carlo Caracciolo queste qualità le possedeva tutte. La ringrazio di avermi dato la parola.

seduta di oggi sia un momento alto di questa Assemblea (tranne qualche stonatura, che perdoniamo perché non merita di essere replicata), che mi rende orgoglioso di appartenervi. Dall'una e dall'altra parte dell'emiciclo celebriamo lo stesso personaggio: commemoriamo Carlo Caracciolo. Lo commemoriamo proprio per la sua capacità umana di essere al di sopra della fazione e della settarietà. Mi permetto, in pochi minuti, di ricordare quarant'annidi amicizia che mi hanno legato a lui. Lo incontrai quarant'anni fa in Germania, ad Hannover, per accordi editoriali; stringemmo e li volemmo celebrare in un momento conviviale, in una cornice non proprio eccelsa, il ristorante della stazione di Hannover, mangiando assieme un terribile *knödel*.

«Sono stato partigiano» ed io dissi: «Io non avevo l'età, sennò sarei stato nelle Brigate nere». Caracciolo mi disse: «Questo non conta: conta la contrapposizione ideale, soltanto quella, senza settarietà, senza faziosità». Ecco, proprio l'opposto di quel senatore che poc'anzi ha dimostrato come si possa essere stupidamente settari, ma forse gli è servito per dargli una qualche visibilità.

senza che fosse da me richiesto, una mattina, dinanzi ad un'aggressione becera, in una canea cretina che forse ha determinato la mia fortuna elettorale,

Sempre, durante la sua vita, io e Carlo Caracciolo ci siamo confrontati in civiltà, con una contrapposizione ideale, ma comunque nella certezza che lui era maestro di dignità umana e di sensibilità. *(Applausi

Nella seduta pomeridiana di oggi, con eventuale prosieguo nella seduta antimeridiana di domani, sarà discusso il decreto-legge sul disagio abitativo, già approvato dalla Camera dei deputati. A conclusione di tale provvedimento, si procederà all'esame del disegno di legge collegato recante delega in materia di produttività del lavoro pubblico. Per il voto finale è richiesta la presenza del numero legale. Nel corso di questa settimana saranno inoltre esaminate le mozioni sulla pirateria in Somalia e sull'integrazione scolastica dei minori stranieri, nonché - ove modificati dalla Camera dei deputati - i decreti-legge già approvati dal Senato in materia di autotrasporto e agricoltura di imminente scadenza e, inoltre, il disegno di legge di ratifica del Trattato di Prum. I lavori della settimana corrente si concluderanno con la seduta pomeridiana di giovedì 18 dicembre, per la quale non è previsto l'orario di chiusura. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi lunedì 22 dicembre, alle ore 11 e alle ore 16, nonché se necessario nella mattina di martedì 23, per la discussione del decreto-legge sull'emergenza rifiuti in Campania, degli altri decreti-legge e argomenti eventualmente non conclusi e inoltre della ratifica del Trattato dì adesione alla NATO di Albania e Croazia, ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati. Dopo la sospensione per le ferie natalizie, le Commissioni potranno riconvocarsi a partire da mercoledì 7 gennaio 2009. I lavori dell'Assemblea riprenderanno martedì 13 gennaio, alle ore 17, con all'ordine del giorno il disegno di legge collegato in materia di federalismo fiscale, ove concluso dalle Commissioni riunite. La ripartizione dei tempi per la discussione di tale provvedimento, l'ulteriore *iter*, nonché la definizione degli altri argomenti da inserire nel calendario alla ripresa dei lavori (tra cui il decreto-legge recante misure anticrisi, documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e il seguito del disegno di legge in materia di sicurezza) saranno stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo nella riunione che sarà convocata martedì 13 gennaio.

Colleghi senatori, il provvedimento in esame è volto a ridurre il disagio abitativo di particolari categorie sociali di conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio nei Comuni capoluogo di Provincia e nei Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, nonché, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ad affrontare, sia pure parzialmente, il tema dei mutuatari insolventi. A tal fine, l'articolo 1 del provvedimento in esame sospende, per un periodo di oltre otto mesi (fino al 30 giugno 2009), la procedura esecutiva di sfratto, limitatamente ai Comuni individuati dell'articolo 1, della legge n. 9 del 2007. Si tratta dei Comuni capoluogo di Provincia, dei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti o ad alta tensione abitativa. Si ricorda che il testo originario prevedeva, invece, la limitazione ai Comuni capoluogo di 14 aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste) ed ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Il blocco delle procedure esecutive di sfratto riguarda i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, aventi i seguenti requisiti: un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro; essere o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata Nello stesso articolo 1 del decreto-legge in esame si precisa che la finalità del provvedimento di sospensione è quella di ridurre il disagio abitativo per tali categorie disagiate in attesa della realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (il cosiddetto Piano casa), introdotto con l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Sotto tale luce, il provvedimento non deve essere inteso come un ulteriore intervento di differimento di termini, bensì come una «sospensione necessaria» affinché sia dato avvio all'effettiva realizzazione del citato Piano casa, che dovrà favorire l'accesso ad un'abitazione in locazione o in proprietà anche per le suddette categorie sociali. Merita qui ricordare che il Piano amplia la platea dei beneficiari includendovi, per la prima volta, gli immigrati regolari a basso reddito e gli studenti fuori sede, finora destinatari, questi ultimi, di agevolazioni di carattere fiscale sui canoni di locazione. La platea risulterebbe ampliata anche dall'inclusione, con un riferimento con un riferimento generico, di tutti i soggetti «sottoposti a procedure esecutive di rilascio». Il comma 1-*bis* dell'articolo 1 prevede che i bandi per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, siano emanati annualmente entro il 30 settembre. Il comma 1-*ter* dell'articolo 1 stabilisce che la sospensione dei provvedimenti di rilascio non comprende i provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore nei casi previsti dall'articolo 3 della legge n. 431 del 1998, tra i quali si ricorda: l'intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, l'intenzione di destinare l'immobile all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, culturali o di culto, qualora sia offerto al conduttore altro immobile idoneo; la piena disponibilità del conduttore di un alloggio libero nello stesso Comune; il grave danneggiamento dell'edificio in cui si trova l'immobile. Il comma 2 dell'articolo 1 dispone invece che, fino alla scadenza del termine del 30 giugno 2009, continueranno a trovare applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, recanti norme di semplificazione e di agevolazione per i conduttori, nonché i benefici fiscali dell'articolo 2 della stessa legge n. 9 del 2007. I benefici fiscali trovano applicazione limitatamente ai Comuni capoluogo di 14 aree metropolitane e ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Il comma 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, che vengono stimate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze può adottare eventuali provvedimenti correttivi nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del decreto, vengano a verificarsi spostamenti dalle previsioni di spesa indicate nel decreto Il comma 4-*bis* incide sull'abrogazione del regio decreto n. 1165 del 1938, Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, disponendo che non vengano però abrogati gli articoli da 118 a 138, come attualmente previsto, ma solo quelli da 118 a 124. Rimarrebbero così in vigore, contrariamente a quanto attualmente previsto dall'articolo «taglia-leggi», le disposizioni che attengono ai poteri del Ministro dei lavori pubblici in materia e prevedono poteri di controllo, di scioglimento e di nomina commissariale. Le disposizioni riguardano anche la commissione di vigilanza, di nomina ministeriale, che ha poteri decisori in materia di graduatorie, poteri sanzionatori e consultivi. L'articolo 1-*bis* introduce l'obbligo, ai fini della valutazione per le graduatorie di edilizia residenziale pubblica, che i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione riportino i dati relativi alla registrazione del contratto e alla lettera di disdetta della locazione. Inoltre, l'articolo 1-*ter* aggiunge, sentite le Regioni, ai fondi già previsti per la realizzazione del cosiddetto Piano casa le risorse del Fondo per l'edilizia a canone speciale, previsto dall'articolo 3, comma 108, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Infine, l'articolo 1-*quater* prevede che gli immobili sottoposti a procedure esecutive o concorsuali, aventi le caratteristiche di quelli di edilizia residenziale pubblica e occupati da mutuatari insolventi, possano essere acquistati dagli Istituti autonomi per le case popolari che stipulano contratti di locazione sostenibili con i mutuatari. La finalità dell'articolo è duplice: favorire la riduzione del disagio abitativo e ridurre le passività delle banche. L'acquisto da parte degli IACP degli immobili, che debbono avere le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed essere l'abitazione principale del mutuatario è previsto senza oneri per lo Stato e quindi con fondi degli enti stessi, che tuttavia possono usufruire delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa. Le locazioni dovranno avvenire secondo canoni sostenibili, il cui importo viene fissato dal provvedimento in esame al 70 per cento del canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998. Si prevede inoltre che esso non sia comunque inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica stabilito in ogni Regione e Provincia autonoma con propria legge. Il canone sostenibile è calcolato come restituzione parziale di quanto pagato per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori dagli Istituti autonomi case popolari. Lo stesso comma 3 dell'articolo 1-*quater* stabilisce che resta ferma la possibilità da parte del mutuatario insolvente, alla scadenza del contratto di locazione, e secondo quanto previsto dalle leggi regionali

Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel nostro Paese la presenza di un'emergenza casa è un dato strutturale. essa rischia di assumere un carattere particolarmente grave a causa delle conseguenze della crisi finanziaria, che comprime, specialmente nei settori sociali più deboli, le possibilità di affrontarla.

soprattutto (e oltre i contenuti) perché i tempi, stanti così le cose, non lo permettono. Per risolvere l'emergenza abitativa, oltre gli interventi a medio termine, occorrono soluzioni nuove, che, a partire anche dalle difficoltà che questa crisi sta evidenziando giorno dopo giorno, siano in grado di avviare e sostenere un percorso articolato che interagisca con un profondo rinnovamento di tutto il sistema Paese. Se le generazioni più anziane difficilmente potranno essere conquistate a prospettive più flessibili di lavoro, dobbiamo convincere le nuove che alla domanda di lavori flessibili, che alla disponibilità di mobilità geografica corrispondono la facilità a spostarsi, a cambiare casa, a trovare servizi adeguati e soprattutto procedure semplici, rapide, economiche ed efficaci. Non è facile allo stato attuale, direi quasi impossibile. Tuttavia l'emergenza va affrontata il rinvio degli sfratti rappresenta nell'immediato una risposta indispensabile soprattutto per le categorie sociali più deboli. Ma il giugno del 2009 purtroppo viene presto e sappiamo tutti che il rischio è quello di ritrovarci a quella data in una situazione poco dissimile dall'attuale. Vorrei prendere spunto dal provvedimento che stiamo discutendo per fare alcune considerazioni più generali. Nel 2006 il 73,3 per cento delle famiglie residenti e il 74,7 per cento degli individui viveva in abitazioni di proprietà.

il rimanente 17,7 per cento di famiglie era in affitto. Oggi in Italia la percentuale delle famiglie proprietarie della casa in cui vivono si può ritenere sia prossima all'80 La percentuale di proprietari è una delle più alte - se non la più alta - d'Europa ed è ovviamente il contrario per gli affittuari. Per capire, almeno quantitativamente, questo elemento nel contesto europeo, come dato estremo di confronto si può considerare la Svizzera, che ha solo il 34,6 per cento di inquilini proprietari delle abitazioni in cui vivono. I dati ai quali faccio riferimento - di fonte ISTAT - sono soprattutto dati che dovrebbero farci riflettere sul sistema Italia, su come affrontare in futuro le politiche per la casa, sul significato e sui modi di affrontare le emergenze abitative e su come tale situazione, pur presentando aspetti positivi, rischi di interagire negativamente aggravando gli effetti La distribuzione della proprietà della casa conferma la percezione che si ha del sistema Italia. Da un punto di vista territoriale, la quota di famiglie proprietarie è più elevata, e in aumento, nel Nord e ancor più nel Centro, dove corrispondentemente si registra anche il calo più consistente nella quota di affittuari. È invece in diminuzione, e inferiore di quasi cinque punti percentuali, nel Mezzogiorno, dove sono però cresciute le famiglie beneficiane dell'alloggio a titolo d'usufrutto o uso gratuito. E' evidente che la fortissima percentuale di case in proprietà delinea una società fortemente statica ed insicura, che ha scarsa fiducia nei sistema Paese e che considera l'acquisto della casa come unico consistente bene rifugio e il cambio di abitazione come un'onerosissima avventura. Ed è altrettanto evidente che sarà sempre difficilissimo parlare di flessibilità specialmente con i giovani - se non si inverte questa tendenza con interventi che sappiano incidere profondamente nella logica del mercato delle abitazioni e negli affitti, riuscendo ad ispirare quella fiducia verso opportunità diverse dall'acquisto che ora non possono esistere. La situazione attuale, tra l'altro, ha contribuito nel tempo a far lievitare i costi delle abitazioni, ha indebitato in maniera consistente le famiglie essendo costrette al ricorso massiccio dei mutui. Un ricorso che inevitabilmente condiziona le stesse capacità di spesa delle famiglie, tanto più in momenti di grave difficoltà come quelli della crisi attuale. L'aumento dei costi, la scarsa disponibilità di abitazioni libere, il prevalere di opportunità stagionali nei molti luoghi turistici, ma, in questo contesto così contorto, anche le difficoltà a rientrare nella disponibilità del proprio appartamento, hanno poi alimentato una crescita continua e a a dismisura degli affitti, crescita che ha colpito tutti, in particolar modo le giovani coppie e, spesso in maniera drammatica, i ceti più deboli. Questa situazione, alle lunghe, ha anche generato uno stato di emergenza permanente, che grava, direttamente o indirettamente e in misura diversa, su tantissime famiglie, in particolare su quelle meno abbienti o che vivono situazioni sociosanitarie particolarmente difficili o gravi. È dunque con questa emergenza che siamo costretti da anni ed anni a continuare a fare i conti.

si è cioè ritenuto, nonostante la conclamata emergenza, di ridurre il numero delle famiglie che, pur nella stessa situazione, ne potessero beneficiare. Stessa tipologia critica d'utenti, stesso problema, ma incomprensibilmente chi non abitava in prossimità di un grande insediamento urbano - anche se in una città a forte densità abitativa - veniva escluso.

Vorrei poi dire che manca in questo decreto l'opportunità di attuare un riequilibrio territoriale del nostro Paese. Siamo una straordinaria penisola, con una

che consentano in generale di recuperare questo rapporto fra centro e periferia attraverso gli enti locali. È opportuno un riequilibrio, anche dal punto di vista costituzionale

*(PD)*. Signora Presidente, l'intervento previsto dal decreto-legge in fase di conversione costituisce un atto responsabile verso una situazione certamente ripetitiva, ma non per questo meno drammatica. Reputo positiva l'estensione della proroga anche a tutti i Comuni ad alta tensione abitativa (secondo la deliberazione CIPE del 2003), che ha risolto una palese diseguaglianza di trattamento fra residenti in Comuni diversi. Oltre a questo intervento estensivo, la Camera dei deputati ha ampiamente modificato il testo originario del decreto-legge. Alcuni emendamenti sono connessi alla proroga, alcuni si riferiscono al reperimento di nuovi alloggi, attraverso il Piano casa ovvero gli Istituti autonomi case popolari. In questo modo, la questione degli sfratti viene, a mio avviso correttamente, inquadrata nel più ampio tema della garanzia dell'abitazione. Occorre una più convinta operatività per il cosiddetto Piano casa, in modo da accelerare la costruzione o comunque l'acquisizione di alloggi popolari. In effetti, la soluzione al problema della dotazione di una casa anche per le famiglie con minore reddito o con conclamate situazioni di disagio costituisce la via maestra anche per una corretta tutela dei diritti dei proprietari, che si trovano sostanzialmente coinvolti nelle procedure di sfratto, che percentualmente sono sempre più connesse alla morosità. L'emergenza abitativa dovrebbe essere affrontata con dati sempre aggiornati (i dati relativi agli sfratti esposti nella relazione tecnica al decreto sono piuttosto arretrati): esistono soggetti istituzionali centrali e periferici, esistono associazioni dell'inquilinato e della proprietà in grado di fornire dati costantemente incrociabili, per un monitoraggio della situazione degli sfratti, sia per finita locazione, sia per morosità. A tal fine abbiamo anche presentato un ordine del giorno. Il tema della morosità non viene toccato dal decreto di proroga, che si riferisce ai provvedimenti di rilascio per finita locazione riguardanti categorie sociali caratterizzate da specifici requisiti. Ma l'analisi delle cause di sfratto evidenzia un aumento dei provvedimenti emessi per morosità e una progressiva diminuzione di quelli emessi per finita locazione. L'effetto del cosiddetto caro-affitti incide sui redditi di fasce sempre più ampie della popolazione, compresa quella zona grigia che non ha un reddito così basso da poter accedere all'edilizia popolare o convenzionata e, nello stesso tempo, non è neppure in grado di acquistare l'alloggio. Sono sperimentabili, in questo senso, anche forme innovative di supporto alle famiglie che affrontano il mercato dell'affitto. Anche in questa prospettiva abbiamo presentato un ulteriore ordine del giorno. Gli amministratori pubblici locali vivono direttamente le spesso drammatiche condizioni nelle quali si risolvono le procedure di sfratto: due interessi importanti e legittimi sono a confronto. Vittime delle situazioni sono soprattutto le persone anziane, quelle in stato di disagio e i minori; sono proprio le condizioni, assieme al limite di reddito, previste per questa proroga. Ogni sfratto eseguito impegna gli amministratori locali, soprattutto nei Comuni medi e piccoli, ad ogni sforzo per risolvere questioni di assistenza sociale non sempre rimediabili. Per questo, mentre è positiva la valutazione per questa ulteriore proroga, sia pure molto definita per tipologia e tempi, sottolineo ancora, in conclusione, la necessità di uno sguardo politicamente più ampio, a sistema, perché la casa sia un obiettivo serenamente perseguibile per tutte le famiglie italiane, con azioni ed interventi significativi ed integrati dello Stato e degli enti locali.

di questo provvedimento. Io vorrei evidenziare alcuni aspetti, se mi è permesso, anche perché ritengo che sia questo il momento particolare per affrontarli. Circa un mese fa - lo

Perché un convegno del genere? Esso ha poi dato vita ad un comitato spontaneo, nel quale sono sono intervenuti l'Ordine degli ingegneri, la Federlazio, l'ACER, l'Assocasa, l'ARPE, l'UGL, la UIL, la CISL e tante altre organizzazioni. Queste ultime, però, sono

sotto l'egida del suo segretario generale, che è Massimo Anderson, e del suo presidente, che è l'avvocato ed ex senatore della Repubblica Michele Pazienza, tanti piccoli proprietari che

e abitazioni per i quali i cittadini fortunati pagano due lire, mentre altri addirittura, caro relatore, non hanno mai pagato niente; e poi c'è chi, in funzione di questo, approfitta

relativa alla costituzione di un comitato promotore degli stati generali dell'edilizia, dove non vi siano solo i rappresentanti dei costruttori (che più non hanno costruito in questo senso),

Roma si parla di 100.000 appartamenti necessari per venire incontro a questi problemi. Un economista quale Fabio Verna parla della realizzazione delle cubature di edilizia sociale, che vanno stabilite, difese e garantite dalla legge; parla della necessità sociale di un intervento concreto dei Comuni in questa direzione, i quali non possono essere abbandonati da soli a trovare soluzione al problema. Marco Di Cosimo, che è presidente della commissione urbanistica del Comune di Roma, nella sua relazione, parla della necessità di reperire ulteriori spazi per la realizzazione di nuovi quartieri, ma io, quando penso ai nuovi quartieri, ho sempre paura che vi sia qualcuno che abbia la volontà di costruire quartieri come Corviale, che sono l'indecenza di un marxismo imperante nell'edilizia degli anni Settanta. *(Applausi del senatore

di entrare in città. È quello un edificio dove tutti sono uguali agli altri, ma nessuno ha l'autonomia della propria abitazione. Quando si costruiscono quartieri dormitorio

coloro i quali su questo argomento hanno i numeri, la possibilità ma anche l'interesse di confrontarsi per aprire un dialogo concreto.

Immagino che sia uno di quegli atti che spesso votiamo, ma di cui in molti faremmo volentieri a meno. D'altro canto, come si può votare volentieri la conversione

Il punto è stabilire se il Parlamento - ma, se volete, lo stesso Paese - possa e debba rassegnarsi ogni anno a prorogare gli sfratti, oppure se continui ad avere un senso interrogarsi e provare a declinare concretamente il diritto ad una casa per tutti.

e a proroghe di sfratto che abbiamo votato negli anni passati. Ci troviamo di fronte ad un'industria delle costruzioni e ad un mercato immobiliare che negli anni sono stati sempre più orientati, dalla politica dei mutui bancari e dalla vantaggiosità di tali investimenti, alla costruzione di alloggi destinati alla vendita. Non mi soffermo sugli svantaggi ambientali e sui costi connessi a certa politica espansiva che ha consumato territorio, magari anche solo al fine di fare cassa per gli enti locali soffocati dai continui tagli centrali; mi interessa di più sottolineare la differenza di questa proroga, una differenza che intercetta la fase economica, le trasformazioni sociali e demografiche e la stessa precarietà lavorativa, che ha ampliato enormemente

senza superare i confini dei diritti di proprietà dei privati, che non possono e non devono essere gli unici soggetti a doversi far carico delle conseguenze derivanti dalla mancanza di una politica abitativa delle istituzioni.

Solo nel 2007 sembra siano state emesse circa 44.000 sentenze di sfratto, di cui circa 34.000 per morosità, sulla quale, come è già stato sottolineato, non si interviene con questo decreto.

Trovo, però, alquanto singolare che, mentre discutiamo di federalismo (quotidianamente ormai), non si introducano norme più stringenti per premiare gli enti virtuosi. Non capisco perché non si analizza quali interventi le Regioni ed altri enti locali stiano realizzando sulla questione dell'emergenza casa.

Ci aspettiamo che maggioranza e Governo affrontino concretamente la questione dell'edilizia abitativa all'interno dei provvedimenti anticrisi, così come ci aspettiamo che l'impressionante aumento del dato relativo agli sfratti per morosità sia assunto ed affrontato negli stessi provvedimenti. In fondo, le due cose sono intimamente legate, non fosse altro che per la constatazione che l'aumento degli sfratti per morosità altro non è che un effetto sociale di una crisi che, per ironia della sorte, ha individuato i primi

colleghi, signor Sottosegretario, altri colleghi del mio Gruppo hanno illustrato le ragioni per le quali il Partito Democratico considera questo decreto come un atto necessario, dovuto, complessivamente condivisibile anche alla luce di alcune modifiche apportate alla Camera con il contributo dell'opposizione, ma come un atto largamente insufficiente a fronteggiare l'emergenza abitativa nel nostro Paese, tanto più nella condizione di disagio socio-economico crescente che vivono centinaia di migliaia di famiglie. Io mi soffermo brevemente su un punto che, ahimè, resta sullo sfondo del decreto che ci accingiamo a votare e sullo sfondo delle politiche del Governo in questa materia. Come ha stabilito la stessa Corte costituzionale, è insensato continuare con la pratica delle proroghe periodiche e sistematiche degli sfratti senza intervenire per dare al Paese risposte sostanziali, strutturali, capaci di fronteggiare la domanda insoddisfatta di *housing* sociale. Nelle città italiane, in particolare, l'offerta di case in affitto a canoni sociali è di gran lunga al di sotto del 10 per cento (4,3 per cento a Roma, 7,2 per cento a Milano), contro una media delle principali città europee vicina al 15 Questo dato così abnorme è in parte il risultato della maggiore propensione degli italiani all'acquisto della casa di abitazione: sia a Roma che a Milano - per rimanere ai due esempi principali di città italiane - oltre il 60 per cento degli appartamenti è abitato dai loro proprietari. È consuetudine presentare tale situazione come una virtù del nostro Paese, e in qualche misura essa certamente lo è. Ma proprio questa vocazione «proprietaria» del mercato immobiliare italiano ha fatto trascurare la necessità di abitare in affitto di una parte comunque significativa del nostro popolo. La mancanza di un'offerta adeguata di *housing* sociale, e soprattutto di case in affitto a prezzi agevolati, è un grande problema per tante famiglie a basso reddito, per le giovani coppie, per gli immigrati, per i giovani che vorrebbero rendersi indipendenti dalle proprie famiglie. Ed è anche un grande problema ambientale, perché alimenta la domanda di case in acquisto a basso prezzo, costruite sempre più lontano dai centri urbani, secondo standard energetici scadenti e al costo di un consumo del tutto eccessivo di suolo. Anche in questo, come nel campo dell'abusivismo edilizio, l'Italia in Europa è un'anomalia. Nel nostro Paese si continua a costruire moltissimo: secondo il rilevamento satellitare condotto nell'ambito del progetto europeo Corine Land Cover 2000,

A Milano, dove negli ultimi decenni la popolazione è diminuita, tra il 1950 e il 1990 l'area urbanizzata è più che raddoppiata (da 114,5 a 233,4 chilometri quadrati, su un territorio comunale di 325,2 sempre a Milano nel periodo 1995-2002 la media annua delle nuove cubature autorizzate è stata superiore ai 30 milioni di metri cubi, contro i 22 milioni di metri cubi autorizzati in media ogni anno nel decennio 1958-1967, cioè all'apice del *boom* edilizio. In Italia si costruisce molto, moltissimo, anche perché per i Comuni gli oneri di urbanizzazione sono tra le principali fonti di finanziamento: ma questo, mentre produce un impatto notevole sull'ambiente e il territorio, non risolve e non ha risolto affatto il fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti. Il Governo, pochi mesi fa, ha annunciato in pompa magna un Piano casa per costruire in due anni 20.000 alloggi. A parte la tempistica del tutto irrealistica, come sa bene chiunque abbia una qualche esperienza di edilizia pubblica o convenzionata; a parte l'impronta fortemente centralistica delle procedure proposte, che escludono i Comuni, gli enti locali dalle scelte su dove, quanto e come costruire; a parte il fatto che ad oggi il piano casa non è che uno dei tanti annunci fatti dal nostro Governo; a parte tutto questo, restano alcune banali osservazioni che consegno in conclusione alla riflessione e al giudizio di tutti i colleghi: per fronteggiare l'emergenza abitativa serve soprattutto costruire case da dare in affitto a prezzi sociali; serve mettere mano dopo oltre mezzo secolo a una nuova legge urbanistica che consenta ai Comuni e in generale alla collettività di acquisire suoli a basso costo per la città «pubblica»; serve riformare la fiscalità comunale che oggi quasi costringe molti Comuni a costruire sempre di più a prescindere dall'utilità sociale del nuovo costruito. Inoltre, ogni piano massiccio di nuove edificazioni deve porsi come obiettivo la minimizzazione del consumo di suolo libero e l'adozione di *standard* elevati di qualità edilizia, energetica, anche estetica per le nuove case. Fuori da questa cornice, il fantomatico Piano casa annunciato dal Governo o rimarrà lettera morta, oppure si tradurrà soltanto in un regalo a pochi grandi speculatori, con danni ingenti per il territorio e senza alcun sollievo per chi vive una condizione spesso drammatica di disagio abitativo. E noi, tra qualche mese, ci troveremo di nuovo a discutere di una proroga degli sfratti. Signora Presidente, onorevoli colleghi, io credo sia giusto e necessario intervenire con un decreto-legge per affrontare la situazione di emergenza casa che costituisce un problema reale, avvertibile in questo momento nel nostro Paese e che, come tale, deve essere affrontato con la dovuta priorità. Il diritto all'abitazione costituisce un diritto sociale fondamentale e l'attuale crisi economica, finanziaria e sociale rischia di minare questo principio. Pensiamo a quante famiglie hanno visto svanire, ancora una volta, il sogno di poter acquistare una casa a causa della recessione di cui oggi siamo tutti vittima, che ha provocato un sovraccarico di interessi e di ulteriori aggravi familiari che hanno contribuito a rendere impossibile la sostenibilità di un mutuo o particolarmente difficile e gravosa la corresponsione di un canone di locazione. Nell'ottica di ridurre il disagio abitativo, penso sia assolutamente ragionevole la decisione della Camera dei deputati di prevedere che gli istituti autonomi case popolari (IACP) provvedano a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari insolventi che occupano gli alloggi. In considerazione della grave crisi dei mutui che ha indotto il Governo a varare ben due decreti-legge a favore delle banche e un altro decreto per accogliere le difficoltà dei mutuatari, occorre vigilare affinché tale disposizione non si traduca in un onere per gli IACP e in un vantaggio invece per le banche, che in futuro non dovranno neppure impegnarsi ad affrontare tutte le procedure di messa all'asta. Dobbiamo prendere atto che la nostra società sta cambiando e c'è una crescente richiesta di case proveniente dai nuovi nuclei monofamiliari. Pensiamo all'aumento dei divorzi, delle separazioni e agli studenti che vivono fuori sede, che rendono necessaria una maggiore disponibilità di alloggi. Ci troviamo dinanzi ad una crescente domanda a fronte di una ridotta offerta di abitazioni, dovuta anche alla dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti previdenziali. Alla luce di queste considerazioni, ritengo opportuna ed avveduta la decisione approvata dalla Camera dei deputati di sospendere per un periodo di oltre otto mesi (fino al 30 giugno 2009) la procedura esecutiva di sfratto nei confronti dei conduttori in condizioni di particolare disagio, abitanti nei Comuni capoluoghi di Provincia e nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, o ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003. Si è così ragionevolmente ampliato l'ambito applicativo del decreto in esame, che limitava il provvedimento di sospensione ai 14 Comuni capoluogo delle aree metropolitane ed ai Comuni ad alta tensione abitativa con esse confinanti. Ritengo sia opportuno segnalare come il provvedimento di sospensione debba essere inteso non come un mero intervento di differimento di termini, ma come una sospensione necessaria affinché sia dato concreto avvio alla effettiva realizzazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, il cosiddetto Piano casa, che dovrà favorire, coinvolgendo soprattutto risorse private oltre a quelle pubbliche, l'accesso ad una abitazione in locazione o proprietà per le categorie sociali più disagiate individuate all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007 e per gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari a basso reddito, categorie purtroppo lasciate fuori dal decreto in discussione e per la prima volta indicate quali beneficiarie. Ai fini della predisposizione delle graduatorie di edilizia residenziale pubblica e dei relativi criteri di valutazione, considerata la penuria di appartamenti disponibili, l'introduzione, fortemente voluta dal Gruppo dell'Italia dei Valori, nel decreto di che trattasi, dell'obbligo che i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione riportino i dati relativi alla registrazione del contratto e alla lettera di disdetta della locazione. Occorre però precisare che, nonostante l'ampliamento di applicazione voluto dalla Camera, il decreto-legge non è particolarmente efficace: secondo noi, si rendono sempre più necessari interventi strutturali nel settore delle locazioni. Ecco perché è sempre più urgente che sia data quanto prima attuazione al Piano casa (che era prevista entro il 5 ottobre 2008), così garantendo su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana. umana. Ci aspettiamo quindi un sollecito intervento del Governo affinché assuma tutte le opportune iniziative per il pronto e auspicato raggiungimento dell'intesa con le Regioni per l'adozione del citato Piano casa. Ma come sempre dobbiamo rivolgere il nostro sguardo alle risorse disponibili. Il Governo dovrebbe darci qualche spiegazione: infatti, ancora una volta intende far fronte alle spese con il Fondo per interventi strutturali di politica economica, già pesantemente tagliato dal disegno di legge finanziaria attualmente in discussione alla Camera e già utilizzato per la copertura dei decreti-legge relativi all'Alitalia, al sistema giudiziario e alle missioni internazionali. Nonostante gli ennesimi tagli e la mancata realizzazione del Piano casa, che riconosce il carattere strategico per il Paese della riqualificazione urbana, che coinvolge, oltre alle risorse pubbliche, quelle private, attraverso il ricorso a modelli di intervento limitati, fino ad oggi, al settore delle opere pubbliche (il cosiddetto *project fìnancing*), e dell'acquisizione o costruzione di immobili per l'edilizia residenziale (il cosiddetto *social housing*), ritengo di poter affermare che la conversione in legge

Abbiamo parti della città che sono dei mostri ecologici per il riscaldamento:

la casa era data sempre ad una certa parte della società; adesso ci si vuole organizzare per vedere di dare la casa agli immigrati, ma dobbiamo tenere bene aperti gli occhi su questa situazione. Quanto ai nostri pensionati,

circolo? Penso che l'Istituto autonomo case popolari per una certa fascia sociale deve pensare di costruire case al sole, non nella nebbia o al freddo della Padania.

dei mostri romani; ne abbiamo anche noi di mostri e mi viene da maledire gli architetti che negli anni Settanta sono riusciti a fare diventare brutte

e come tale appare in continuità rispetto ai provvedimenti meramente emergenziali che si sono succeduti in questi anni. Ricordo che su provvedimenti di questo tipo vi fu una battaglia proprio al Senato da parte di esponenti del Gruppo del PdL nel 2006, con l'approvazione da parte dell'Assemblea di una pregiudiziale di costituzionalità, presentata dai colleghi Pastore e Ferrara. In realtà, questo provvedimento è strutturalmente diverso rispetto al passato, perché riduce le ipotesi in cui opera la proroga, le limita all'accertamento dei meri casi di bisogno e riconosce anche il bisogno del locatore, la sua necessità di di poter disporre per sé o per i propri figli della abitazione data in locazione. Vi sono provvedimenti innovativi che consentono a chi

finalmente la predisposizione finalmente di una azione del Governo, di una nuova politica, anticipata con un provvedimento presentato immediatamente con l'entrata in Il Piano casa presenta meccanismi innovativi ed intelligenti, che hanno lo scopo di aggredire finalmente la problematica, non limitandosi a governarne l'emergenza; meccanismi premiali ai diritti edificatori per chi realizza interventi residenziali nei quali inserisce alloggi di edilizia pubblica o di edilizia convenzionata, valorizzazione del ruolo dei promotori, costituzione di fondi dedicati ad investimenti in alloggi che devono poi essere posti sul mercato a prezzi calmierati, riavvio del programma di dismissione dell'edilizia residenziale pubblica. È quindi un contesto nuovo quello nel quale si inserisce questo provvedimento, che in tal senso assume

bisogna vedere cosa è accaduto negli ultimi dieci anni, per vedere come si è sbagliato e quali sono le prospettive sulle quali l'azione del Governo ci ha oggi condotto. La crisi del sistema di edilizia pubblica si avvia con l'abolizione da parte del Governo Prodi del prelievo GESCAL. Da allora non sono mai state più

Negli anni 2000 vi è stato il boicottaggio delle Regioni e degli Enti locali, in particolare di quelle di centrosinistra, che impugnarono financo gli atti governativi davanti alla Corte costituzionale sul primo grande piano di dismissioni dismissioni avviato dal Governo Berlusconi, che prevedeva il diritto e la possibilità dei conduttori, degli assegnatari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di acquisirlo ad un prezzo calmierato. Badate bene, rispetto al dibattito in Aula, dobbiamo significare la nostra azione rivolta verso il soddisfacimento del diritto alla casa, anche e soprattutto riconoscendo non solo al quasi 80 per cento degli italiani, ma alla totalità delle delle famiglie italiane la possibilità di acquisire una casa di proprietà nella quale vivere. Ma su questi temi vi è stata per anni una politica contro la casa e contro la proprietà della stessa, caratterizzata da una presenza forte della sinistra massimalista anche nei rami parlamentari, che è stata per anni condizionante della politica del Governo. All'ostilità con cui si è riusciti a fermare il piano di dismissione dell'edilizia residenziale pubblica, che avrebbe consentito da una parte ad assegnatari di diventare proprietari e quindi soddisfare per sempre il loro diritto e d'altra parte di reperire risorse che avrebbero potuto potuto costituire una base importante, vorrei dire quasi imponente, per rilanciare altre azioni a favore di chi aspetta e non vedeva soddisfatto il proprio bisogno, si è aggiunta anche una serie di norme, soprattutto a livello regionale, con le quali si sono estesi a dismisura i criteri di accesso alle graduatorie di edilizia pubblica. È vero quanto diceva il collega Leoni, che sul tema dell'edilizia residenziale pubblica si è totalmente perso in molte Regioni l'intento di qualificare e riconoscere il diritto di cittadinanza. il diritto di cittadinanza. Per esempio, nella mia Regione, l'accesso alle case di edilizia residenziale pubblica è oggi unicamente riservato agli abitanti delle nostre città, non cittadini italiani e non residenti, che spesso si trovano in una fascia di emarginazione superiore.

poter entrare nelle graduatorie e comunque ha privilegiato tutte le forme di convivenza diverse da quella fondata sul matrimonio. Questi sono dati di fatto che il Governo ha ben presente, che abbiamo denunciato in questi mesi e che rappresentano un tema sul quale non possiamo tacere. Così come non possiamo tacere gli eccessi di un ambientalismo di maniera, che ha impedito il rinnovamento delle città ed ha preteso di ingessare il nostro territorio, comportando in alcune realtà una grandissima crescita del valore dei beni immobiliari, connessa ad una maggiore domanda rispetto all'offerta del mercato.

il soddisfacimento di un bisogno pubblico senza preoccuparsi dei problemi o dei bisogni che gli stessi avevano. Non dimentichiamo poi che la politica della proroga degli sfratti, andando a incidere sui contratti liberamente assunti, ha portato progressivamente nelle grandi città a sottrarre al mercato degli affitti una quota importante del patrimonio immobiliare. La politica delle proroghe, a fronte a fronte della necessità di avere garanzie per il futuro in merito alla disponibilità dei propri beni, ha portato anche alla riduzione degli alloggi che potevano essere affittati, perché lo Stato non ha in questi anni garantito che i contratti venissero onorati e che il diritto alla proprietà della locazione potesse avere la propria pienezza. Quindi, anche su questo tema, e concludo, respiriamo un clima diverso e nuovo. nel sostenere questo provvedimento, presentiamo anche un ordine del giorno volto a rafforzare la necessità di attuare questa nuova politica ed interventi strutturali. Con esso si chiede anche al Governo un impegno affinché la politica della proroga degli sfratti indiscriminata, che abbiamo conosciuto nel passato e che già oggi è

del sistema delle autonomie, insieme a quello dello Stato, possa produrre i risultati che, ahimè, nel recente passato non ci sono stati, qualche volta anche per colpevole volontà da parte delle amministrazioni regionali.

non toglie che sia un bene molto caro per milioni di persone. Forse non era così qualche anno fa, negli anni Settanta e fino a metà degli anni Ottanta, quando si costruivano con l'aiuto dello Stato circa 30.000 alloggi

È inutile dire che in questi anni i vari Governi che si sono succeduti non hanno voluto affrontare la questione della casa. Oggi questa opportunità non c'è più. Non si può minimamente pensare che una Nazione civile, alle soglie delle terzo Il progresso è altra cosa per il centrodestra: la società, come il centro-destra la pensa e l'ha disegnata, è cosa diversa. Il welfare deve necessariamente L'obiettivo è quello di sintetizzare le caratteristiche complessive del modello italiano, di una politica pubblica nel settore immobiliare, di discutere di eventuali proposte di riforma anche alla luce delle esperienze straniere e degli orientamenti dell'Unione europea, dell'Unione europea, che rappresenta un attore sempre più importante e principale nei processi interni di politica economica e sociale. Tutti i settori di intervento pubblico devono fare i conti con vincoli o opportunità collegate al nuovo livello di governo sovranazionale. In molti paesi Europei il diritto ad una abitazione decente fa parte a pieno titolo della cittadinanza sociale. quale motivo in questi anni non si è mai pensato ad un fatto del genere in Italia. Nel nostro Paese la politica della casa è rimasta sempre ai margini della politica sociale, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello puramente simbolico. Per noi la casa è il posto in cui vivere. Pensare ad una politica per la casa significa pensare anche devono sviluppare le nostre città e gli spazi della vita privata in relazione alla vita associativa. La casa è una vera e propria realtà culturale: rappresenta l'identità dei paesi, delle città, dei territori e dei popoli.

economia familiare, la casa è qualità della vita, è cultura, la casa è estetica, è etica; la casa è il futuro della nostra società, la casa è il tempo libero, è la qualità del lavoro, è la qualità della vita, è la politica. Dobbiamo rapportarci a tutto questo per costruire un'Italia migliore. Questo provvedimento è stato reso necessario dagli eventi e dal poco tempo che abbiamo avuto a disposizione. Esso rappresenta senz'altro l'inizio di una nuova stagione politica per la casa; era nei nostri programmi e siamo intenzionati a mantenere

Ho ascoltato tutti gli interventi che sono stati svolti, a cominciare dalla senatrice Granaiola che ha parlato di tema emergenziale della casa,

I Comuni hanno già dato il proprio assenso, contrariamente alla posizione delle Regioni. L'ANCI ha già dato infatti la propria disponibilità a trattare sul tema della casa; le Regioni, invece, in questo momento pongono ancora qualche difficoltà, che sono certo sarà superata.

per quanto riguarda in particolare la registrazione dei contratti e il tema della disdetta, che certamente per noi è importante. Sul tema della casa visto che parliamo di un patrimonio pubblico, ci deve essere il rigore necessario per qualsiasi intervento si debba adottare. Al senatore Leoni, che ringrazio per il colorito intervento, ricordo che, pur abitando anch'io nella Pianura Padana,

in maniera che ogni città ha costruito in proprio, realizzando quelle periferie cui il senatore Leoni ha fatto cenno. Effettivamente, è importante

della distribuzione dei fondi, così com'è avvenuta finora, sia comunque da osservare. Allora, si è ritenuto di far intervenire

il senatore che mi ha pregato di intervenire volesse dirmi se posso concludere, lo farei volentieri, visto che mi sembra di parlare per nessuno.

è certamente riferito alle famiglie a basso reddito, alle giovani coppie a basso reddito, alle categorie svantaggiate, agli studenti fuori sede, alle famiglie soggette a procedure di rilascio e agli immigrati che sono residenti da almeno dieci anni in Italia e da cinque anni nella Regione. Va detto che per quanto riguarda la situazione attuale, le Regioni dispongono di fondi ex GESCAL - come riferito dalla Cassa depositi e prestiti - di 1.560.000.000 di euro che sono ancora disponibili e non impegnati. Questo deve spingerci a far capire alle Regioni che è indispensabile ed opportuno sedersi ad un tavolo per poter far partire davvero questo piano casa. Visto che vi è stata richiesta, sia alla Camera che al Senato, di un dibattito pieno sul tema della casa, è chiaro che il Governo è a completa disposizione per soddisfare tali richieste.

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che, in relazione alle procedure di cui all'articolo l-*quater*, si tratti di una mera facoltà degli enti, posta in essere soltanto compatibilmente con l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e soltanto per le situazioni di insolvenza già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,

e morosità, che raffronti i dati certi e certificati a disposizione dei soggetti istituzionali centrali e periferici e delle rappresentanze degli inquilini e della proprietà».

Siccome c'è anche un scolaresca in Aula è bene dare l'esempio. Ho già detto che c'è una richiesta di rigore ancora maggiore. Rivolgo un invito alla responsabilità di ogni singolo senatore chiedendo, al contempo, ai colleghi senatori Segretari di

In premessa ci si deve rammaricare del fatto che l'esame degli emendamenti al Senato è stato condizionato da tempi ristretti dovuti all'imminente scadenza del decreto, per evitare la quale, pur presentandoli, abbiamo rinunciato alla loro illustrazione inoltre che sia mancata la possibilità di disporre, prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, del parere della Commissione bilancio, che è stato comunicato a inizio seduta. I nostri emendamenti sono volti a migliorare il testo del provvedimento in alcuni aspetti principali, tenendo conto dell'impossibilità tecnica di restituire il provvedimento alla Camera. In particolare, riteniamo che il Governo debba impegnarsi a concedere più detrazioni fiscali per i proprietari che affittano a canoni ragionevoli come efficace disincentivo agli affitti in nero; chiediamo l'avvio di politiche che consentano anche ai lavoratori precari l'accesso ai mutui o alle locazioni. Proponiamo inoltre l'impegno a realizzare, a partire dal Piano casa che deve essere celermente avviato, misure che agevolino direttamente le famiglie, anche monoparentali o monoreddito, nonché interventi volti a bloccare temporaneamente le procedure esecutive concorsuali qualora l'inadempienza di un mutuatario non sia dovuta a colpa, negligenza o malafede. Abbiamo chiesto altresì un monitoraggio sistematico della situazione del patrimonio abitativo pubblico, per reprimere gli abusi che vi si registrano diffusamente a spese degli aventi diritto, e una seria analisi del mercato immobiliare delle locazioni, in modo da potere assumere a ragione veduta decisioni simili a quelle che altri Paesi europei hanno preso da anni. Ricordiamo infine la nostra perplessità, di metodo ancor prima che di merito, sull'articolo 1-*quater* e sulle modifiche riguardanti il Testo unico sull'edilizia popolare Alcuni ordini del giorno incidevano anche sugli articoli in questione, richiamando, in conclusione, la necessità di un più attento esame dei parametri soggettivi ed oggettivi cui possono corrispondere in futuro eventuali provvedimenti dotati di incisività, ma il Governo ha espresso

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se ho ben capito visto l'andamento della discussione, mi verrà chiesto di ritirare l'emendamento e valuterò cosa fare, ma non rinuncio ad una sobria illustrazione. In Commissione affari costituzionali ci siamo trovati assolutamente d'accordo su tre questioni: che sussistessero i requisiti di necessità ed urgenza; ed urgenza; che si trattasse di problematiche di tale rilievo e delicatezza di ordine sociale, specialmente in questo momento di difficoltà per tante fasce sociali della nostra Nazione, questione è che probabilmente non stiamo rispettando i canoni costituzionali rigorosi riguardo alle pari opportunità, a diritti ed aspettative dei cittadini residenti nelle varie località, nei vari Comuni e nei vari territori. territori. Il provvedimento, infatti, aveva preso le mosse, come da impulso del Governo, per un'emergenza abitativa in alcune poche metropoli, sicuramente contrassegnate - specie in alcune zone e quartieri - da un'effettiva emergenza abitativa, mentre i nostri colleghi parlamentari della Camera hanno ritenuto opportuno allargare la previsione di questo intervento a tutti i Comuni capoluogo di Provincia e a quelli - badate bene - con essi confinanti. Si tratta di mezza Italia, signori colleghi, per cui si discrimina automaticamente l'altra metà del Paese. Ci siamo trovati d'accordo - ed una mia osservazione al riguardo ha trovato autorevoli appoggi, come quello del senatore Pastore, per la maggioranza, o del senatore Ceccanti, per l'opposizione - nel dire che il principio, il criterio, il parametro del capoluogo di Provincia non può più trovare ingresso nei provvedimenti legislativi che vanno a stabilire insediamenti, articolazioni dello Stato sul territorio, interventi finanziari: in questo modo, non solo si accentuano gli squilibri, che non sono giustificati, ma anzi, si va contro la tendenza maggioritaria del Parlamento e delle forze politiche, oltre che - se permettete - del programma di Governo della coalizione della quale mi onoro di far parte, di superare l'istituto della Provincia e della sua dimensione territoriale. A questo punto, per tali considerazioni, abbiamo detto vieppiù che è inconsistente questa divisione tra capoluoghi di Provincia e non in materia di edilizia abitativa e di emergenza.

tra la città di Termoli e quelle di Isernia o Campobasso. Tutto ciò è assolutamente fuori dalla logica e dal raziocinio; è anzi spesso vero il contrario. Preannuncio quindi il ritiro dell'emendamento, perché la questione è di tale rilevanza e delicatezza sociale che non mi sento evidentemente di contrastare un provvedimento del genere; ma mi incoraggia soprattutto il fatto

che impegna l'Esecutivo a non produrre più e a non dare più attuazione a provvedimenti che abbiano come parametro istituzionale territoriale discriminante quello del capoluogo di Provincia.

anche se so che non saranno approvati per la decisione della maggioranza di difendere il testo, così come è uscito dalla Camera dei deputati, perché cercano signor Presidente, richiamo anche la sua attenzione perché temo che di questa norma sentiremo ancora parlare - di precisare l'ambito di applicazione della norma contenuta nell'articolo 1-*quater*, che a mio giudizio è una vera e propria enormità. Vorrei che fosse chiaro che cosa stiamo votando e cosa contiene questa norma: si riferisce al soggetto che ha fatto un mutuo ed è attualmente proprietario di una casa su cui vi è l'ipoteca relativa allo stesso mutuo, che non ha pagato le rate e ha la casa sottoposta a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale. Ebbene, in questo caso, purché la casa non sia di categoria catastale A1 e A2, cioé una casa di grandissimo lusso, dice la norma è possibile che un ente pubblico, l'Istituto autonomo case popolari o come si chiama adesso - non è importante - interviene e compra la casa. Fin qui si dice che è un

Il canone sociale che viene pagato non va però all'Istituto autonomo case popolari, ma alla banca che aveva erogato il mutuo e l'istituto case popolari, cioè un soggetto pubblico, ci mette la differenza fino ad arrivare al concorso dell'intero canone di mutuo. Una volta fatto questo, alla fine, l'Istituto autonomo case popolari arriverà naturalmente a pagare l'intero mutuo, nel frattempo si sarà fatto carico dei costi di manutenzione della casa e così via

La norma non contiene, signor Presidente, alcun riferimento alle condizioni sociali in cui si deve trovare la famiglia (ecco perché l'emendamento in questione

perché non prevede una data di riferimento che sia tale, per cui l'intervento è a valere su condizioni che si sono già determinate nel passato. Potremmo avere un Enrico Morando che abita in un tale Comune e che decide adesso di non pagare più la rata del mutuo e poi si mette a brigare per fare in modo che l'Istituto autonomo case popolari paghi per suo conto la rata del mutuo, salvo, tra dieci anni, ricomprarsi la casa da capo. Ma ci rendiamo conto di quali sono le conseguenze in termini di trattamento delle persone per bene in questo Paese, di coloro che sputano sangue ma poi alla fine la rata del mutuo la pagano?

si fissano per legge le condizioni di *status* e di reddito alle quali le famiglie devono rispondere per poter beneficiare di tale intervento e si stabilisce che le famiglie in questione pagheranno almeno la quota

l'imbarazzo dei colleghi della maggioranza e del Governo nel dichiarare che una norma del genere non comporta oneri per la finanza pubblica è evidente dal parere della

Se il Governo accettasse di introdurre almeno una data dopo la quale tale procedura non sia più attivabile, norma, riferendosi la stessa solo a casi che si sono aperti nel passato. Ma l'idea di lasciare aperta la norma per i casi che si determineranno nel futuro, signor Presidente, è veramente imbarazzante. Finisco dicendo: attenzione, se qualche istituto autonomo case popolari si metterà a fare questa operazione, nel giro di sei mesi spenderà tutti i soldi che deve utilizzare per costruire le case popolari ai poveracci.

senatore Morando ha colto l'occasione dei due precedenti emendamenti per introdurre un argomento già sollevato dal Gruppo del Partito Democratico all'interno della discussione svoltasi in Commissione ed emerso in numerosi interventi svolti in Aula. È chiaro che qui siamo di fronte a un problema:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1260, impegna il Governo a far sì che, conformemente alle finalità perseguite con il decreto-legge 20 la disciplina recata dall'articolo 1-*quater* del medesimo decreto-legge trovi applicazione con riferimento ai soli soggetti appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 1 del decreto-legge e alle sole situazioni determinatesi anteriormente all'entrata in vigore legge di conversione». È infatti di tutta evidenza che l'articolo 1-*quater*, così come è scritto, si presta ad un'interpretazione estensiva; esso non è collegato immediatamente ai fruitori del decreto in questione,

della norma in questione ai soli soggetti che vivono situazioni determinatesi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto e, nello stesso tempo, alle sole categorie sociali cui fa riferimento l'articolo 1. Colgo l'occasione per

Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo parlamentare UDC, SVP e Autonomie

ed ha diritto, come tutti gli altri che seguiranno, al silenzio.

Intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole sul provvedimento in esame, anche se riteniamo che la risposta fornita sia insufficiente a contenere il disagio abitativo

Sottolineo, in merito al Piano casa, che questa era l'occasione per destinare parte dei fondi che sono stati recuperati nel decreto‑legge in esame per dare una risposta anche a migliaia di famiglie che non riescono più a pagare il mutuo. Era necessario intervenire in questo settore destinandovi magari quei 30 milioni di euro già stanziati per tale finalità dal Governo Prodi e per i quali Tremonti aveva confermato l'impegno in questo senso. Sottolineo, tra l'altro, che stiamo parlando di sfratti che riguardano solo particolari categorie sociali. Voglio ricordare al Governo che la maggior parte degli sfratti nel nostro Paese non si riferisce solo alla fine della locazione, ma soprattutto alla morosità, il che testimonia la gravità della situazione economica. Il Piano casa che è stato annunciato deve dare una risposta possibilmente organica al settore, soprattutto sul piano sociale, ma direi anche dal punto di vista economico. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione, non prima di aver sottolineato un aspetto che viene trascurato. Per quanto riguarda i 16 miliardi di euro per le infrastrutture, perché

Così sulla casa daremmo una risposta sul piano sociale, ma soprattutto manterremmo in moto lo sviluppo dell'economia, rilanciando le piccole e medie imprese, perché sulla casa lavorano ben 32 settori produttivi. Oggi, per il dramma che nel Paese si vive nelle grandi aree urbane, la risposta non può che essere positiva per rilanciare l'edilizia residenziale pubblica che da troppi anni non trova un'adeguata risposta. Se il Governo riuscisse a fare questo, probabilmente non parleremmo più di proroghe, ma daremmo una risposta definitiva per questo settore.

Il voto del Gruppo Italia dei Valori del Senato sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo sarà favorevole. Tuttavia, riteniamo doveroso sottolineare come i dieci giorni scarsi concessi al Senato per esaminare il decreto non abbiano consentito ai parlamentari che siedono in questo ramo del Parlamento, siano essi di maggioranza come di opposizione, di far valere una serie di osservazioni, a volte anche critiche ma più spesso finalizzate ad apportare aggiustamenti e modifiche migliorative, né di approfondire con la dovuta riserva di tempo un tema delicato come quello della crisi delle politiche abitative. Il copione che prevede la marginalizzazione del Senato si ripete questa settimana con il decreto per l'emergenza rifiuti in Campania, che già ci arriva blindato. Il primo effetto importante che si produce è certo quello di dare breve respiro agli inquilini. Ma dobbiamo qui constatare come, man mano che i decreti di blocco si rinnovano, la platea dei beneficiari venga sempre più riducendosi, fino alle poche migliaia di unità attuali, come evidenziano i dati della nota di lettura del Servizio bilancio del Senato. Nella Relazione tecnica si stima, in base a dati di fonte ministeriale, un numero totale di provvedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione emessi annualmente pari a 9.838, mentre gli sfratti bloccati risulterebbero pari a 2.889. Resta evidente la necessità di una inversione della dinamica distorta dei prezzi immobiliari come sistema per far tornare il bene casa accessibile ai cittadini con reddito medio, come accadeva fino a pochi anni fa, a meno di non volerli indurre ad indebitarsi ulteriormente e ad incappare negli inconvenienti che la crisi dei mutui ha portato all'attenzione di tutti e anche del Governo, il quale è dovuto intervenire con un decreto che prevede addirittura la garanzia dello Stato, a carico dei contribuenti quindi, su mutui contratti da privati cittadini qualora superino un dato livello (fissato però in modo che le odierne dinamiche dei tassi lo renderanno con ogni probabilità irraggiungibile).

Come ho detto in discussione generale, mi auguro che quanto prima il Senato della Repubblica esamini un disegno di legge per la casa.

tale rottamazione potrebbe fungere proprio da motorino di avviamento per il rilancio dell'economia. Su questo vi sono meravigliosi esempi: esempi: penso a Barcellona, dove, in occasione delle Olimpiadi del 1992, gli architetti (quelli giusti) hanno ridisegnato la città.

un patrimonio di edilizia sociale pari a 4,5 abitazioni ogni cento. I Paesi Bassi avevano nel medesimo anno

a dimostrare, ancora una volta, come siamo distanti dall'Europa, ma soprattutto come siamo distanti dall'aver affrontato questo problema non solo in chiave di emergenza, ma in chiave di risoluzione stabile, di ricerca di risposte vere ai problemi veri della gente. Ancora. Che cos'è il problema dell'affitto in Italia? In Italia, alla fine degli anni Settanta, inizio anni Ottanta, poco più del 20 per cento degli affittuari era in condizione di povertà.

Alla fine degli anni Settanta e all'inizio degli anni Ottanta, per circa il 60 per cento degli affittuari il peso del canone di locazione non superava il 10 per cento del reddito disponibile; negli anni 2000, il 45 per cento dei nuclei in affitto si vede togliere, per pagare i canoni di locazione, almeno un quarto del reddito disponibile. Capite che di fronte a questi dati non c'è solo la questione dell'emergenza sfratti per le categorie

esca dalla pura declamazione, dalla pura indicazione verbale e diventi qualcosa di concreto per il nostro Paese. Ovviamente il Piano casa suppone molte cose, innanzitutto che venga ridata centralità agli enti locali. Noi non siamo per un Piano casa che veda solo il Governo e gli organismi centrali decidere, allocare risorse e prendere decisioni sui grandi progetti di sviluppo abitativo. Vogliamo un coinvolgimento serio degli enti locali, vogliamo che il ruolo dei Comuni sia valorizzato. E ancora. Come possiamo affrontare un Piano casa se, come già è stato detto in interventi autorevoli che mi hanno preceduta, non facciamo una riflessione seria sull'utilizzo delle aree in questo Paese? Il Piano casa deve anche prevedere, a mio modo per non consumare ulteriormente le aree che abbiamo e quindi riutilizzare aree dismesse e mal edificate in anni lontani ed oggi non più utilizzabili in modo serio ai fini residenziali. Vuol dire affrontare il problema del risparmio energetico delle nostre abitazioni, affrontare il tema dell'architettura sostenibile e della bioarchitettura. È chiaro, quindi, che un Piano casa non deve meramente andare in una direzione; non si deve solo edificare tanto per edificare, ma occorre tener conto della domanda di qualità e di sostenibilità ambientale che in questi anni è è cresciuta ed è diventata, fortunatamente, patrimonio di molti. Ancora. Credo che dobbiamo capire che c'è un mercato che riguarda l'affitto, ma c'è anche un mercato di case che devono essere rese fruibili per una platea di cittadini a reddito medio (giovani coppie, ad esempio) che hanno bisogno magari sui tempi lunghi, a poco a poco, di poter acquisire la casa come

proprio nell'imminenza della sua decadenza per decorso dei termini. Non so fino a quando le Commissioni e l'Aula del Senato riusciranno a reggere

come è stato fatto anche nel corso del dibattito, l'esigenza, nell'interesse dei provvedimenti, di promuovere alcune modifiche. La seconda considerazione, sempre di carattere procedurale, ma anche sostanziale, è relativa all'articolo 1-*quater*. Nel corso del dibattito alla Camera, per iniziativa di più parti politiche, non certo della nostra,

Abbiamo cercato di ovviare con un chiarimento interpretativo del quale penso il Governo vorrà fare immediato tesoro, ma forse sarebbe stato più opportuno stralciare interamente

il fatto che il Governo, tra le sue prime iniziative, abbia assunto quella di varare un nuovo Piano casa e siamo certi che lo farà nei tempi necessari perché questo decreto non abbia bisogno di essere reiterato. Questo è un impegno che il Governo ha assunto: il Parlamento lo recepisce e la maggioranza attende con ansia e soprattutto con grande disponibilità il provvedimento sul Piano casa, che sicuramente, dopo tanti decenni, com'è stato detto in quest'Aula, segnerà una nuova politica di

di prime case private nel contesto europeo. Occorre cioè considerare una connotazione del nostro tessuto sociale che, come si suol dire in gergo, è molto legato al mattone sicuramente alle politiche abitative della prima casa. Infatti, nel nostro Paese sempre tanti sono stati, ad opera di più Governi anche di vario indirizzo politico, gli interventi a favore dell'acquisto della prima casa, soprattutto in occasione della formazione di nuove famiglie o a vantaggio delle famiglie disagiate. Ancora una volta apprezziamo che il Governo abbiaimmediatamente focalizzato uno dei problemi fondamentali

ripeto - alla prassi dei provvedimenti di proroga continua, che determinano incertezza del diritto e anche una certa conflittualità sociale. quindi certo che nei prossimi mesi, affrontando il problema del Piano casa, porremo le basi per una vera, nuova e strutturale politica abitativa nel nostro Paese. Ringrazio tutti i componenti della Commissione

Signor Presidente, non ho voluto interromperla durante la sua ottima conduzione dei lavori dell'Assemblea, ma vorrei avere semplicemente due chiarimenti. Ella ha giustamente ricordato che in Consiglio di Presidenza il presidente Schifani ha raccomandato la correttezza nell'utilizzo delle tessere;

richiesta di porre in discussione la mozione sulla situazione economica internazionale. Mi permetto di sottolineare che,

un ulteriore aggravamento della crisi economica e finanziaria internazionale, che potrebbe rendere ancora più urgente l'espressione di un'opinione e di indicazioni da parte dell'Aula